Onorevoli colleghi, il Consiglio di Presidenza si è riunito ai sensi degli articoli 12 e 67 del Regolamento con riferimento ai fatti accaduti nel corso della seduta dell'Assemblea del 15 giugno 2017. Il Consiglio ha udito i senatori coinvolti che ne hanno fatto richiesta e riscontrato i Resoconti e i video relativi alla seduta, assumendo le seguenti determinazioni. Il Consiglio deplora in modo fermo tutte le condotte poste in essere dai senatori che hanno turbato l'ordine dei lavori e assunto atteggiamenti e usi di linguaggio censurabili verso l'istituzione, la Presidenza e un Capogruppo della Camera dei deputati. Per tali ragioni, sono state irrogate all'unanimità, con effetto immediato, le seguenti sanzioni, ai sensi dell'articolo 67 del Regolamento del Senato, nei confronti dei senatori: Calderoli e Volpi, la censura; Arrigoni, Consiglio, Crosio, Divina e Tosato la censura e l'interdizione di partecipare ai lavori del Senato per un giorno di seduta; Centinaio la censura e l'interdizione di partecipare ai lavori del Senato per due giorni di seduta.

sono emersi senza alcun dubbio vari problemi: al di là delle criticità del contenuto - quello è un altro aspetto - sono emersi problemi di carattere tecnico a proposito della copertura.

Grazie

Grazie

poi non è colpa mia se in Parlamento sono stato audito perfino sulle mense scolastiche, ma nessuno ha pensato di chiamare il Presidente dell'ANAC quando si stava per fare una modifica devastante» - riferendosi a quella introdotta dal codice antimafia - «che ammazzerà le misure di prevenzione. Non sono solo io a dirlo ma pure Canzio» (che, per chi non lo sapesse, è il primo Presidente della Corte di cassazione), «Fiandaca» (noto giurista), «Cassese» (notissimo principe del diritto italiano, professore, già membro della Corte), «Flick» (già Presidente della Corte), «Rossi, De Lucia. Siamo forse diventati tutti pazzi?». Così dice Cantone.

ci consente, nelle forme dovute, di realizzare un codice antimafia più forte. Signor Presidente, lo dico con molta serietà. Nel 1999 ero già parlamentare - ahimè, credo che questo oggi sia

sono fonti qualificate ed esperte, quanto le nostre. Ognuno di noi, Presidente, pur non essendo stato procuratore o altro, ha dato un contributo alla legislazione del Paese, nel senso di una maggiore severità nei confronti delle cosche e delle organizzazioni criminali.

Io sono contrario all'inversione proposta dal senatore Malan, perché sono curioso di vedere come va a finire il codice antimafia. È dall'inizio che sono curioso di vedere come finisce. Quello che è avvenuto ieri è un fatto di assoluta gravità; ci siamo legati mani e piedi da soli. Dopo le ultime tre dichiarazioni di voto, arriveremo ad affrontare il famoso coordinamento finale obbligatorio; annuncio già da ora, Presidente, che ritenendo che quel coordinamento non sia tale, perché non armonizza alcunché in contrasto con l'articolo 32, ma va invece ad esplicitare quello che non c'è scritto in tale articolo - che, ricordo, è stato già votato due volte - chiederò una convocazione della Giunta per il Regolamento, al fine di verificare se quel coordinamento sia ammissibile, se sia un coordinamento o non sia, in realtà, un emendamento mascherato. Francamente, fossi stato uno dei relatori, avrei presentato un emendamento con un articolo aggiuntivo, in cui si andasse a specificare ed esplicitare che i 20 milioni stanziati per l'articolo 32 erano

ma certamente le modifiche al codice antimafia al nostro esame avrebbero avuto bisogno di parecchi perfezionamenti. Intanto, avrebbero avuto bisogno di una maggioranza e di un'opposizione che si fossero parlate e ascoltate, ma così non è stato. Poi avrebbero avuto bisogno di un maggiore coordinamento tra gli Uffici legislativi di Camera e Senato e si sarebbero probabilmente evitati errori materiali marchiani, cui la Commissione giustizia ha cercato come ha potuto di porre rimedio, e si sarebbe forse evitata anche la scena, che non si è ancora conclusa, di un coordinamento finale, per dare risposta all'obiezione della Commissione bilancio sulla copertura Naturalmente questo coordinamento avrebbe comodamente potuto e dovuto trasformarsi in un emendamento, in Commissione o in Aula. C'è poi dell'altro e lo voglio dire con franchezza, dandone dandone atto ai colleghi parlamentari della destra, che ne parlano spesso. In quasi tutti i provvedimenti che arrivano dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati e che passano per le mani della sua Presidenza c'è una tendenza che definirei pericolosa, che a me sembra quella

è stato sviato da "armi di distrazione di massa", come la riforma costituzionale, che è stata poi bocciata clamorosamente dalla grande maggioranza degli italiani, e quella elettorale, cassata dalla Consulta.

siano stati considerati dalla nostra maggioranza di Governo come i canditi nella cassata siciliana, che sono un po' un condimento barocco, a beneficio dell'immagine e della vista, mentre la la sostanza della cassata è la crema di ricotta che c'è all'interno. Così si fa un pessimo servizio alle istituzioni e si rischia di paralizzare il Parlamento in una lotta senza costrutto.

cari senatori, non credo, caro Presidente. Ho la sensazione che la vera ragione di questa forte ostilità è che le modifiche al codice antimafia colpiscono i reati contro la pubblica amministrazione e la corruzione. Sono reati di cui in Italia sono quasi sempre responsabili i galantuomini, le personalità politiche o i soggetti che con tali personalità hanno rapporti. si tratta di soggetti che, nel nostro Paese, molto raramente finiscono in carcere, a differenza di Paesi come la Germania o gli Stati Uniti, che spesso amiamo portare ad esempio. Oggi, a protezione dell'impunità di persone che sono spesso responsabili di un pesante danno alla vita economica e democratica del Paese, dovremmo dunque bloccare il provvedimento? Penso che non possiamo farlo. farlo. I colleghi della destra chiedono perché si sia voluto intervenire con il sequestro preventivo dei capitali di cui non si può spiegare l'origine,

La risposta è quella che diede Aureliano Buendía: «*Hoc est simplicissimum*»: la mafia, infatti, vede nei reati contro la pubblica amministrazione e la corruzione dei reati ancillari.

dell'uomo considereranno oggi il patrimonio come un'estensione consustanziale della persona umana e, quindi, dei suoi diritti inalienabili. Il punto fondamentale è che se c'è un'emergenza mafia, noi dobbiamo sapere che c'è una fortissima emergenza corruzione. vi dicevo di Reggio Calabria e Trapani, ma se voi andaste a Palermo - cosa che vi invito a fare - avreste la sensazione che la mafia non ha più il "fiato" su quella città.

economia e società lavora solo, o quasi esclusivamente, di commesse pubbliche, dove la corruzione è il sale del contratto fra corrotto e corruttore, tra imprenditore che vuole per forza l'appalto e politico che lo vuole dare perché così può dimostrare

Ogni volta che si parla dei nostri martiri si sprecano gli elogi, ma temo che li si dimentichi nella realtà. Senatori, quasi cinquant'anni fa è toccato anche a me, allora giovinotto, di scrivere delle cose che al tempo sembravano bizzarre. Scrissi che la mafia non era soltanto *killer* ma principalmente era intermediazione. L'immagine era quella del Giano bifronte, con un volto rivolto al potere romano e un volto che era inutile mandare i mafiosi al confino e che bisognava colpirli nel patrimonio, nella «roba», perché quello era il punto. Queste posizioni sembravano allora il delirio ideologico di una minoranza più o meno rivoluzionaria non importabile dentro lo Stato di diritto. Mon è stato così,

che ha avuto un magistrato come Chinnici, che fu ucciso per questo. Quando allora ricordiamo le nostre vittime, ricordiamo per che cosa sono morte, perché usare questo tipo di strumenti, avere un'idea della

le dichiarazioni del Presidente del PD sono imbarazzanti e molto preoccupanti. Io ora non parlo di Cantone e non parlo di Flick perché con loro discuteremo. Io penso abbia ragione la presidente Bindi, ma se il provvedimento fosse sbagliato avremo tempo per correggerlo. Parlo però di Orfini: perché Orfini scopre solo ora che quel tipo di provvedimento interdittivo e di sequestro non si può usare nei confronti della corruzione? Perché non l'ha scoperto prima? Chi ha seguito l'*iter* di questo provvedimento? Ho la sensazione, come dicevo prima, che queste leggi siano state trattate come i canditi della famosa cassata siciliana e che oggi vengano inopinatamente a galla, perché non si è interrotta la legislatura e perché le famose riforme sono state un insuccesso, e allora ci si preoccupa soprattutto per ragioni di tipo elettorale ed esiste il rischio

che accada, che dai banchi dell'opposizione e della maggioranza ci fosse uno scatto d'orgoglio e si tentasse di evitare una fine miserabile della legislatura.

condividiamo, a differenza di Forza Italia di altre forze di centrodestra, la necessità e l'urgenza di una riforma del testo unico antimafia. Soprattutto siamo favorevoli, contrariamente al centrodestra, all'estensione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali nei confronti degli indiziati di reati gravissimi come sono quelli della corruzione e della concussione. Per questo motivo abbiamo tenuto un atteggiamento responsabile che ha consentito al provvedimento di arrivare fino a questo punto. Certo, noi lo avremmo scritto in maniera diversa perché rimangono tutt'ora molti punti critici fra

allora, se è accettabile un compromesso al ribasso quando parliamo di mafia e corruzione. Io credo di no. Credo non sia accettabile,

oggi si possono disporre misure di prevenzione quando sussiste l'abitualità delle condotte illecite, la pericolosità sociale del soggetto o quando si ritenga che viva abitualmente dei proventi di attività delittuose. Con la vostra introduzione del vincolo associativo il rischio (di tipo interpretativo) è che queste misure di prevenzione non si possano più applicare se non nei casi, del tutto minoritari e difficili da dimostrare, di corruzione in associazione. Il rischio è dunque quello di un clamoroso autogol, di un passo indietro nel contrasto ai fenomeni corruttivi nel nostro Paese. In altre parole, limitando l'applicazione della norma ai cosiddetti corrotti in associazione, si rischia di escludere l'azione di prevenzione nei confronti di coloro che non delinquono in forma associativa, seppure siano delinquenti abituali di elevata pericolosità sociale che vivono abitualmente dei proventi di attività illecite. Potrebbe così venire impedita persino la confisca dei beni a quei corrotti che, fuori dai circuiti associativi, utilizzassero sistematicamente la corruzione per arricchirsi. Come se non bastasse, la norma che introduce le misure di prevenzione nei reati contro la pubblica amministrazione, a differenza di quanto era stato approvato in Commissione, non trova applicazione nei casi di corruzione dove l'aggravante associativa non c'è o semplicemente non è dimostrabile o non è di facile dimostrazione. A questo punto mi chiedo quale sia stato il ruolo di Berlusconi, di Ghedini, di Gianni Letta relativamente alla stesura del citato emendamento; mi chiedo perché questa modifica non sia stata portata in discussione in Commissione, ma al contrario sia stata scritta in qualche segreta stanza (non si sa bene da chi) Presidente, è stata presentata in Aula una modifica sostanziale al provvedimento all'ultimo minuto, dopo tre anni di discussione dello stesso nelle Aule parlamentari. Insomma, siamo alle solite: in Commissione si concorda un testo efficace per contrastare i fenomeni corruttivi nel nostro Paese, fenomeni che sappiamo benissimo essere terreno fertile per il radicamento della mafia; si porta il provvedimento in Aula forti di un'ampia maggioranza, salvo poi cambiare le carte in tavola e presentare un emendamento che rappresenta indiscutibilmente un compromesso al ribasso, un boccone amaro che vorreste farci ingoiare. Noi in materia di lotta alla corruzione e alla mafia non possiamo e non vogliamo accettare compromessi al ribasso.

un ruolo strategico nella gestione ed amministrazione delle aziende confiscate. Sappiamo tutti che Invitalia è un carrozzone pubblico, i cui dipendenti non sono stati assunti con le garanzie di un concorso pubblico, ma al contrario sono stati scelti dalla politica secondo logiche clientelari. Ebbene, i dipendenti di Invitalia potranno gestire le aziende confiscate economicamente più rilevanti. Capisco benissimo la *ratio* *ratio* alla base di questa norma: consentire la gestione di queste aziende a persone vicine al vostro partito, che siano del PD o di Forza Italia non cambia niente. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Secondo voi questa logica risponde agli interessi dei cittadini?

ma il risultato non cambia) gli emendamenti tesi ad aumentare le tutele per i testimoni di giustizia, creando le premesse per una oggettiva disparità di trattamento. Sono state poi cancellate le modifiche introdotte alla Camera dal Movimento 5 Stelle che prevedevano la possibilità per i poliziotti di ristrutturare e usufruire delle abitazioni confiscate alla mafia e che si trovavano in stato di abbandono. Inoltre, non sono state considerate le conseguenze sul piano della responsabilità in capo agli amministratori giudiziari per il caso di nomina di amministratori che si trovassero in situazioni di incompatibilità o di conflitto d'interesse.

attribuiti questi beni sempre ai soliti soggetti, alle solite cooperative e alle solite organizzazioni. In conclusione, l'abbiamo già visto con il 416-*ter*, una riforma quest'ultima animata da buonissime intenzioni ma sbagliata nella sua formulazione, che ha avuto la conseguenza di liberare dal carcere i condannati per voto di scambio politico-mafioso in primo e in secondo grado. L'abbiamo già visto anche con la riforma delle norme anticorruzione, una riforma fallita, inefficace, solo di facciata, un clamoroso appuntamento perso da questo Parlamento con la storia del nostro Paese. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Ebbene, anche oggi con questo provvedimento, pur riconoscendone e condividendone molti obiettivi, non intendiamo renderci complici dell'ennesimo compromesso al ribasso in materia di contrasto a mafia e corruzione. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Per questo motivo, dichiaro che il voto del Movimento 5 Stelle sarà di astensione.

Signor Presidente, qualcuno in questi giorni si chiede il perché del nostro impegno su questo provvedimento e qualcuno parla di ostruzionismo, ma probabilmente dimentica che il Governo Berlusconi ha introdotto il codice antimafia nel nostro Paese in linea di continuità con le prime norme in materia di antimafia di La Torre,

quello di garantire il sequestro dei beni (la cosiddetta "roba") degli eredi dei mafiosi, quello di aver tolto il gratuito patrocinio agli imputati di mafia per garantirlo alle donne vittime di violenza. Queste sono le regole. C'era allora la necessità di una correzione del codice? Certamente sì.

recepire legislativamente. Secondo aspetto. C'era una gestione corretta dei beni sequestrati alla mafia? No, perché vi era una responsabilità (o non vi era) dei cosiddetti professionisti dell'antimafia. Ce lo siamo chiesti? Quali indagini ha svolto la Commissione Quali indagini ha svolto la Commissione per stabilire se, per ipotesi, nei reati di mafia c'era stata un'attenzione o vi erano delle modifiche normative da apportare? Perché dico questo? un terzo soltanto dei sequestri arriva alla confisca, mentre gli altri due terzi non è che non arrivano a confisca perché passa il tempo, ma perché vengono bocciati vengono eliminati dai successivi processi, che riguardano i sequestri che sono stati disposti. Bisognava anche valutare quali erano gli strumenti perché fosse garantito il rispetto della legalità, da un lato, e la possibilità di utilizzazione dei beni, dall'altro. Eppure avete votato contro

Abbiamo poi avuto la possibilità di discutere, signor Presidente, una serie di torsioni forzature del procedimento legislativo, che pongono in forse la stessa legittimità di questa legge. Ciò porta ad ulteriori conseguenze. Non l'ho detto io: l'ha detto Cantone e l'ha detto Violante. Qual è il problema? Il problema è che aver esteso le misure antimafia anche ai reati contro la pubblica amministrazione può comportare

Il presidente Grasso ricorderà che quando abbiamo fatto il codice antimafia non abbiamo parlato di indiziati per quanto concerneva il terrorismo e il partito fascista; significava un'altra cosa: l'indiziato riguardava la mafia, perché quest'ultima e la corruzione sono due cose diverse. Volete continuare a discutere? Io voglio discutere ancora,

ho rispetto e mi tremano le vene nel momento in cui vedo giuristi di chiara fama che dicono una certa cosa e mi pongo il problema se sia corretto quanto dichiaro. signor Presidente, in quest'Aula ci sono "giuristi" che se ne fregano di quello che hanno detto (non certo

di modificare una norma già approvata. E allora, se per caso doveste fare anche quest'altra cosa assurda,

io mi chiedo: siete proprio convinti che queste norme, così come sono state scritte, serviranno nella lotta alla mafia?

che per interessi personali gestisce in un certo modo i beni sequestrati alla mafia? Noi volevamo dare un'attestazione di ritorno alla legalità, da una parte, con l'attribuzione alle forze di polizia; ma, dall'altra, significava anche riaffermare un principio e dire grazie a chi combatte per la legalità tutti i giorni.

voi non potete introdurre ulteriori allargamenti di sistemi che contraddicono i principi di civiltà giuridica del nostro Paese. E quando qualcuno, pur di

presidente Grasso sa quanto io fossi vicino ai magistrati di Palermo e ciò significa che ancora oggi io credo che la lotta alla mafia vada combattuta con tutti gli strumenti necessari. Proprio per questo,

mafia. Io poi non ho parlato delle torsioni e delle forzature del procedimento legislativo, che già da sole avrebbero giustificato un voto contrario. provvedimento, perché si tratta di una legge che, anziché migliorare quegli strumenti cui noi abbiamo dato la prima attuazione completa,

Presidente, resto convinto che tra poco approveremo un provvedimento importante, che migliorerà l'azione di prevenzione e contrasto alle mafie e la gestione dei beni confiscati. È un provvedimento frutto di un lavoro lungo, che non può essere riassunto con l'articolo 1. Un lavoro lungo, iniziato sui territori, con la presentazione della legge di iniziativa popolare di modifica del codice antimafia, promossa da migliaia di associazioni che oggi ci chiedono di votare il codice in fretta e la cui voce credo abbia la stessa dignità di altre in quest'Aula. proseguito con la presentazione e l'approvazione da parte delle Camere del documento di analisi e proposta prodotto dalla Commissione antimafia. è arrivati alla presentazione e alla approvazione alla Camera di questo disegno di legge, con il voto della maggioranza, della Lega e di altri Gruppi. Un provvedimento che oggi abbiamo ulteriormente migliorato e che potrà tornare a Montecitorio per il sì definitivo. Sono passati trentacinque anni dall'approvazione della legge Rognoni-La Torre, che ha consentito il sequestro preventivo dei patrimoni dei mafiosi, di colpirli lì dove sono più sensibili, restituendo alla collettività ciò che è stato loro sottratto. Quella legge, quell'idea, che qualcuno qui ha definito una follia degna dei regimi del passato, è stata il salto di qualità che ha cambiato la storia della lotta alla mafia e ha consentito di dare colpi durissimi alla criminalità organizzata.

garantire le banche dati, consentire la presenza di personale stabile, qualificato e sufficiente per svolgere le mansioni che gli vengono attribuite, cambiare le procedure di intervento sulle aziende sequestrate per gestire quelle in grado di stare sul mercato, salvaguardando l'occupazione delle persone perbene e liquidando, invece, quelle non in grado di avere un futuro con la delega al Governo della normativa per tutelare i dipendenti. Il codice antimafia interviene sui sequestri giudiziari per evitare abusi e distorsioni, migliorare la capacità di governo delle imprese. C'è molto altro in questo disegno di legge. Ne hanno parlato i relatori e molti colleghi in discussione generale. Quello che voglio sottolineare è che il provvedimento all'esame mette il Paese nelle condizioni di amministrare al meglio e in modo trasparente un patrimonio che, grazie al grande lavoro di magistrati e Forze dell'ordine, diventa sempre più consistente; una ricchezza per l'Italia che va valorizzata e che non possiamo più permetterci di lasciare inutilizzata cosicché si svaluti. La legge Pio La Torre nasce da un'intuizione: colpire i patrimoni con i sequestri preventivi e le confische per contrastare e combattere i reati di mafia. Oggi, contrariamente a quello che è stato detto qui più volte, contrariamente a ciò che Parlamento europeo e molti Paesi europei guardano a quelle stesse misure patrimoniali preventive come a uno strumento indispensabile per la lotta alla criminalità e si propongono di introdurle anche nei loro Paesi, anche con una direttiva europea. Io rispetto tutte le idee, ma l'idea che trova applicazione nel disegno legge - e di cui si è molto parlato in queste ore di usare le stesse misure di prevenzione personali e patrimoniali per i reati gravi contro la pubblica amministrazione non è un'invenzione giustizialista. Significa con la stessa logica prevenire reati odiosi, come la corruzione, che colpiscono la collettività, potendo attivare misure di prevenzione, quelle stesse misure di prevenzione che oggi sono utilizzate non solo per la lotta alla mafia ma - per esempio - per colpire reati come la violenza negli stadi, l'uso della droga e il mancato rispetto del DASPO. Stiamo parlando di misure che per questi reati sono già applicate, e non si capisce perché non debbano essere applicate anche per la corruzione. Certo, non bisogna consentire l'abuso delle norme ma è corretto pensare che sia giusto, attraverso il sequestro preventivo dei beni e dei patrimoni che si ritengano di provenienza illecita e sottratti al pubblico, garantire che vengano restituiti alla collettività alla quale sono stati sottratti, senza che sia possibile occultarli. Tra l'altro, i reati contro la pubblica amministrazione, a partire dalla corruzione, sono spesso segno di una situazione di diffusa illegalità, in cui le mafie si insinuano. Aggiungo anche che l'estensione delle misure di prevenzione al terrorismo - contenuta in questo disegno disegno di legge - è decisiva per contrastare i finanziamenti al terrore. In tema di applicazione delle misure di prevenzione anche per i reati contro la pubblica amministrazione ho sentito in quest'Aula parole forti: rischio di totalitarismo, di regime, attentato ai diritti e alle libertà dei cittadini. Non è così e lo sapete bene. Lo sa bene chi ha usato quelle parole. Altrimenti deve spiegare a quest'Assemblea perché si è arrivati qui senza aver neppure presentato un solo

Occorre dimostrare innanzitutto che il tenore di vita di quelle persone, il patrimonio di quelle persone è molto superiore a quello che potrebbe essere garantito dal loro reddito.

e non si possono sequestrare beni superiori a quelli che si ritiene siano stati sottratti alla collettività. Diciamo la verità. In più, questo provvedimento esce dal Senato migliorato e solo grazie alla maggioranza e ai relatori che, con il loro emendamento, coerente con le osservazioni del procuratore nazionale antimafia, che qualche citazione avrebbe meritato di avere nella discussione svolta *(Applausi dal Gruppo PD)*, hanno tolto il peculato d'uso e chiarito che, oltre all'abitualità, è necessario che ci siano reati associativi

Mi si consenta un accenno anche al tema delle interdittive e dei certificati antimafia, su cui ho ascoltato diversi interventi critici durante la discussione. Quella sulle interdittive è un'altra delle norme che si sono rivelate tra le più efficaci nella lotta alla mafia. Credo che, prima della tutela delle imprese, che credo sia giusta e necessaria, si debba in questa sede prendere atto che le inchieste, da quella in Emilia fino a tutte quelle sulle mafie al Nord, ci parlano del tentativo delle mafie di entrare e insediarsi nell'economia legale e ci raccontano di un'impresa di un'impresa chiusa ogni tre giorni perché infiltrata dalle mafie. Se non partissimo da qui, sembreremmo gente che vive sulla Luna. Valorizziamo invece il fatto che proprio grazie alle interdittive, agli accessi ai cantieri, al lavoro delle prefetture, stiamo contrastando con successo i tentativi della 'ndrangheta e soci di penetrare nelle grandi opere: da Expo (92 interdittive) fino al Giubileo. E di fronte a ciò, è interesse anche delle imprese sane, che non vogliono una concorrenza non libera perché condizionata dalle mafie, non indebolire gli interventi per contrastare le infiltrazioni. Ho già detto che questo provvedimento è importante, modifica il codice antimafia migliorandolo ed aggiornandolo. Altro che indebolire la lotta alla mafia! un altro atto importante contro le mafie che conferma l'impegno di questa maggioranza e di questo Parlamento contro la criminalità organizzata, un impegno che abbiamo dimostrato in questa legislatura. Voglio fare per gli scettici propagandisti un elenco delle misure approvate in quest'Assemblea che hanno dato più forza e più strumenti allo Stato per la lotta alle mafie: la modifica dell'articolo con l'introduzione del voto di scambio (voti in cambio di favori), che dopo tre anni - come conferma ancora la Direzione nazionale antimafia - ha mostrato di produrre risultati positivi; la reintroduzione del falso in bilancio, la cui abolizione aveva chiaramente reso più difficile combattere corruzione e capitali mafiosi; l'introduzione del reato di autoriciclaggio, la legge anticorruzione ed il codice degli appalti.

non è vero quello che dice quella persona, e cioè che la lotta alla mafia in questo Paese si è indebolita. Abbiamo fatto molto; la lotta alla mafia l'abbiamo fatta veramente; il nostro Stato ha le forze, le intelligenze, le competenze per sconfiggere le mafie. La magistratura e le Forze dell'ordine, alle quali va il nostro ringraziamento, sono sempre impegnate e i risultati delle ultime settimane lo confermano: 60 arresti di mafiosi l'altro giorno, 116 arresti di martedì sulla costiera ionica, gli arresti dei capi 'ndrangheta Barbaro a Platì e Giorgi a San Luca. Si è molto parlato del baciamano del *boss*. Ma qui dobbiamo con orgoglio sottolineare l'arresto di due *boss* proprio nei santuari della 'ndrangheta che sembravano inaccessibili per lo Stato. E l'altro giorno un'altra operazione importante, con 116 arresti, proprio in quei territori è stato un segnale forte. Altro che non si fa la lotta alla mafia. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Anche per questo, per confermare con orgoglio il nostro impegno contro le mafie, voteremo a favore del provvedimento in esame e ricordo a me stesso che abbiamo preso l'impegno perché venga approvato in via definitiva al più presto. Questa legge serve, dà strumenti più efficaci per combattere le mafie, valorizza le tante forze civili e sociali che danno un contributo importante per la legalità. E soprattutto dimostra che le istituzioni - il Parlamento in testa - non mollano: guardano come le mafie cambiano, adeguano i mezzi di contrasto e continueranno nei prossimi anni - ne siamo sicuri - a dare colpi sempre più forti alle organizzazioni criminali. Grazie all'opinione di molti colleghi e, a nome del progetto «Energie per l'Italia», annuncio che voterò contro questo provvedimento perché vizia ulteriormente un sistema di giustizia già malato. La speciale possibilità di disporre rilevanti misure cautelari sul patrimonio di persone sole indiziate per reati contro le pubbliche amministrazioni non risulta certo attenuata dall'inserimento del loro carattere associativo. Sono state e sono troppe le indagini temerarie, che ora riguardano anche l'insindacabile attività parlamentare, per non temere l'abuso di misure che produrrebbero danni certi e immediati a fronte di un esito a lungo differito nel tempo, comunque incerto, molto spesso favorevole all'indiziato. Devono rimanere, quindi, speciali gli strumenti di contrasto del crimine organizzato e del terrorismo, mentre devono collocarsi, anzi, in un più effettivo rispetto delle garanzie quelli relativi ai reati ordinari, per quanto socialmente riprovevoli.

Presidente, ho apprezzato le dichiarazioni e gli interventi del senatore Caliendo. Tuttavia, pur trovando fondate le motivazioni per un voto contrario, personalmente non parteciperò al voto, come ho visto faranno anche altri colleghi; ho letto le dichiarazioni Grazie Angelino Alfano, ministro degli affari esteri, ha affermato che il suo Gruppo chiederà robusti cambiamenti al testo alla Camera. Voterete a favore di un testo che il *leader* del vostro partito e del vostro Gruppo definisce da cambiare? Voglio che rimanga agli atti la mia non partecipazione al voto, perché

su «Il Mattino» di Giuseppe Tesauro, già presidente dell'*Antitrust*, della Corte costituzionale e di qualsiasi cosa abbia avuto a che fare con il diritto in Italia: «Il rimedio è peggiore del male», è il titolo del suo articolo. Cito i titoli perché i tempi sono brevi. Boccia,

osservazioni critiche per rafforzare la lotta alla mafia. Pertanto, non partecipo alla votazione su un codice antimafia che aiuta il crimine, smentisce i maestri del diritto, dovrà essere corretto e qui tornerà. Fate un regalo ai corrotti e alla mafia. Io a questo non ci sto.

Signor Presidente, chiedo, se possibile, un minimo di attenzione. Qualche mese fa abbiamo licenziato un disegno di legge in tema di programmazione delle demolizioni dei manufatti abusivi, abusivi, in copia conforme al testo pervenuto dalla Camera, con una sola eccezione: in quel provvedimento c'era scritto che un determinato fondo doveva valere per il triennio 2016-2019. Trovandoci nel 2017, evidentemente la norma meritava una correzione. Si disse all'epoca che non si poteva fare un coordinamento formale

Ah, parlava con lei, bene. Come dicevo, in questo precedente il triennio 2016-2019 non poteva essere oggetto di una modifica in triennio 2017-2020 attraverso il coordinamento formale. Adesso ci viene proposto un coordinamento formale che sostanzialmente tripartisce la somma di 20 milioni per gli anni 2018, 2019 e 2020, secondo le previsioni della Commissione bilancio, che potrebbero ben essere del tutto diverse da quelle che ciascun senatore può immaginare o da quelle che magari, con uno studio più approfondito, potrebbero essere più idonee all'attuazione della delega. È questo un coordinamento formale o una modifica sostanziale? Il problema è tutto qua.

era stato oggetto di un coordinamento formale. E con riferimento a quel coordinamento formale, signor Presidente, leggo che quelle condizioni poste dalla Commissione bilancio - parlo all'epoca della Commissione - recavano «modifiche di carattere sostanziale che avrebbero dovuto essere più opportunamente introdotte attraverso la presentazione di veri e propri emendamenti». Questa non è una mia valutazione, signor Presidente, ma è la sua: è esattamente quello che lei ebbe a dichiarare nella seduta pomeridiana del 21 aggiungendo, per un principio di conservazione degli atti, che, poiché in Commissione non era stata prevista la procedura aggravata e sostanzialmente non vi era una grande differenza tra i coordinamenti della Commissione e i singoli emendamenti, in via del tutto eccezionale si sarebbe potuti andare avanti. Aggiungeva però, signor Presidente, che il carattere eccezionale di quella procedura non poteva e non doveva costituire in alcun modo una prassi:

che sempre ella, signor Presidente, ebbe a dire che, nonostante il carattere del tutto eccezionale della procedura seguita, il procedimento in sede referente si configura più flessibile e meno formalizzato rispetto alle regole della discussione in Assemblea». Orbene, signor Presidente, non credo, alla luce del suo dire, di quello che lei ha affermato il 21 giugno 2017, che la proposta di coordinamento formale, avanzata dalla Commissione bilancio, possa essere considerata un vero e proprio coordinamento formale, apportando delle modifiche a un testo nella tripartizione della somma, peraltro al testo dell'articolo 32 che è stato votato autonomamente, quando si è votato quell'articolo, e che si è votato nuovamente - nonostante quello che il senatore Ferrara ha cercato di spiegare nei suoi interventi - con la votazione dell'articolo 36, e prima dell'emendamento che andava a modificare l'articolo 36, così come ricordato ricordato dal senatore Calderoli. 2017 e dell'obiettiva incidenza di quel coordinamento formale sul merito dell'articolo 32, peraltro votato ben due volte, credo non si possa procedere ad un coordinamento formale.

Presidente, è una ben strana situazione. Ieri il presidente Orfini dichiarato che questo testo sarebbe stato modificato alla Camera, dove si sarebbero fatti carico delle obiezioni che l'Autorità nazionale anticorruzione e diversi insigni giuristi hanno mosso su di esso. Oggi il ministro Orlando afferma che questo testo non deve essere cambiato alla Camera, perché un'eventuale e ulteriore navetta farebbe correre il rischio di una mancata approvazione del provvedimento. Non abbiamo certezza di tipo politico in ordine al futuro. Verrà cambiato o non verrà cambiato;

Qualcosa dobbiamo fare.

essere. Presidente, credo che la proposta non possa essere considerata un coordinamento formale. ogni caso, ove la strada dovesse essere questa, mi associo alla richiesta fatta dal senatore Calderoli, relativa all'immediata convocazione della Giunta per il Regolamento.

con riferimento a delle sue precedenti prese di posizione sulla natura sostanziale di determinati coordinamenti e sul fatto che non sono stati accettati analoghi e meno incisivi coordinamenti formali. Credo, quindi,che la Giunta per il Regolamento debba essere convocata. Poi so bene che nella Giunta per il Regolamento ci sono le maggioranze e le minoranze. Ma, quantomeno, sarà tale Giunta a esprimersi in maniera definitiva su un problema così importante, che tocca un disegno di legge particolarmente delicato e - non nascondiamocelo, perché non lo possiamo fare - che corre il rischio di inficiare l'intera struttura del disegno di legge. intervengo per illustrare la proposta di coordinamento formale, che avevo già preannunciato informalmente ieri, ai sensi del prima comma dell'articolo 103 del Regolamento,

Detto in altre parole, vorremmo togliere l'inciso «del delitto di cui all'articolo 416 del codice penale, finalizzato alla commissione...» con riferimento ai criteri di ammissibilità dell'applicazione delle misure di prevenzione per i reati di corruzione. In parole ancora più semplici, per chi ci dovesse seguire al di fuori di questo palazzo, la nostra più grande preoccupazione, già rappresentata dalla dichiarazione di voto del mio Capogruppo, in relazione all'articolo 1, è che l'aver inserito la settimana scorsa, nel corso la limitazione della contestazione o contestabilità, seppur a livello indiziario, dell'ipotesi associativa, di cui all'articolo 416 del codice penale - si ha quando almeno tre persone si mettono d'accordo per la realizzazione di una serie di reati - sia un criterio che limita in maniera considerevole la possibilità che sequestri e confische per fatti di corruzione possano trovare ingresso nel nostro ordinamento. E dico

oggi permetterebbe alla magistratura di richiedere e applicare misure di prevenzione anche ai reati contro la pubblica amministrazione, questa novella legislativa potrebbe dare adito a una interpretazione secondo la quale un giudice, in futuro, potrebbe sostenere che il legislatore del 2017, avendo indicato come criterio essenziale l'associazione a delinquere per i fatti di corruzione, ha voluto dire che la pericolosità sociale non debba essere più collegata alla reiterazione dei reati, al tenore di vita o al patrimonio superiore a quello dichiarato o a quant'altro. Il criterio a cui fare riferimento deve essere l'ipotesi associativa,

preoccupazione non può essere suffragata da elementi di fatto, perché stiamo parlando di ipotesi e possibili interpretazioni future. Magari ci sbagliamo o magari no, ma nel dubbio vorremmo

di anticorruzione, nella consapevolezza che ciò potrebbe addirittura essere determinante per il voto finale del Gruppo Movimento 5 Stelle. Grazie

avanzata dai banchi del centrodestra, di tornare in Commissione per un momento di approfondimento, al di là di ogni strumentalizzazione politica o parlamentare? al collega Mirabelli, mi spiace doverlo smentire, vista la passione della sua articolata dichiarazione di voto. Vorrei ricordare al collega e a tutti noi che il centrodestra nel suo complesso e, in particolare, i colleghi Sacconi, Di Maggio,

Dicono esattamente quello che lei, oggi, ha provato a negare, e cioè che qua nessuno si è preso la cura di

Questo dissenso mi porta a dire che la delicatezza e la complessità di questo dibattito, che per altro va avanti da parecchio tempo,

che noi stessi contribuiamo a determinare quando alimentiamo continuamente il caravanserraglio della burocrazia:

di aver depositato in data 20 aprile una sua relazione ove è ripetutamente scritto che non è condivisibile la traslazione *tout court* della normativa antimafia alla corruzione. corruzione. Trovo che ciò sia preoccupante per un Governo che deve poter mantenere, nel rapporto con la sua maggioranza e con l'intero Parlamento, la totale correttezza e uno scambio di informazioni che finora abbiamo sempre visto garantiti anche nei provvedimenti e nei momenti più difficili o delicati. Mi riferisco - per esempio - a un provvedimento

che cosa si sta realmente facendo, anche ben oltre quel decreto. Il punto, però, è che questo o l'altro ramo del Parlamento devono assumersi la responsabilità

coscienti, consapevoli e responsabili. Noi, e solo noi.

dei senatori Langella, Malan, Barani, Bernini, D'Anna, Caliendo, Mazzoni, Pagnoncelli Marin e Floris, alcune delle quali identiche tra loro. La proposta di coordinamento presentata dai relatori corrisponde al parere espresso dalla Commissione bilancio. In tale parere la Commissione ha integrato quanto espresso in precedenza, in precedenza, confermando il nullaosta sul testo del provvedimento e condizionandolo, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, ad una specificazione su base annua della copertura di cui all'articolo 32, A questa stregua la proposta di coordinamento dei relatori, analogamente ad altre proposte avanzate da altri senatori, è considerata ammissibile. Viceversa la Presidenza non considera ammissibile la proposta di coordinamento presentata dai senatori Cappelletti e Buccarella, poiché il contenuto è estraneo alla previsione di cui all'articolo 103, comma 1, del Regolamento.

per mettere ai voti una proposta di coordinamento che trae origine dal parere espresso ieri dalla Commissione bilancio. Gli ottimi Uffici sono stati ben attenti ieri, nel momento in cui hanno inoltrato il parere (estensore il che questo fosse scritto in modo molto attento e che quindi citasse al suo interno la parola: «integrazione» e le parole: «deve intendersi». In questo senso, quindi,

che le disposizioni contenute in un disegno di legge che sono contrarie all'articolo 81 della

Cosa succede a questo punto? Noi abbiamo posto ai voti l'articolo 27 e l'articolo 32 con un parere che di fatto, visto che poi è stata introdotta un'integrazione, aveva una sua contrarietà.

Quindi ora come facciamo a coordinare qualcosa che dovrebbe essere espunto, perché è stato votato senza che fosse risolto e che fosse osservata una precisa prescrizione regolamentare, cioè quella dell'espunzione senza il parere? Noi oggi non stiamo coordinando, ma stiamo riportando in vita qualcosa che non dovrebbe esistere. Infatti, in assenza del parere della 5a Commissione o, meglio, essendo il parere della 5a Commissione un parere contrario, l'articolo 32 è *tamquam non esset*. Ora, possiamo fare di tutto e di tutto è stato fatto in quest'Aula. Il senatore Azzollini probabilmente non lo ricorderà nel suo intervento e a questo punto, se mi permette, lo ricordo io. Nelle leggi di bilancio (lo sanno perfettamente gli Uffici quando ne ho parlato ieri, che prevedevano un po' di tutto, modifiche di copertura e quant'altro) mai è successo che una norma di coordinamento, che fosse risolutiva di problemi notevoli, fosse fatta

Quando occorreva questa unanimità, l'allora Presidente della Commissione bilancio senatore Azzollini andava dal collega senatore Morando, si otteneva un accordo, lo si sottoponeva a tutte le parti, si raggiungeva l'unanimità e poi si votava.

la proposta di coordinamento, ci si accordava espungendo, correggendo o dicendo «questo non è possibile», «questo non lo possiamo fare», «no, questo lo si faccia», e lo mettevamo ai voti. stiamo per votare una proposta di coordinamento sulla quale parliamo da due giorni. Il Presidente ha un potere assoluto in quest'Aula, che discende dall'articolo 100 Ma, rispetto al potere assoluto del Presidente, derivantegli dall'articolo 100, c'è anche un potere sovraordinato, quello della legge principale, cioè della Costituzione, e quindi quello dell'osservanza del Regolamento in quanto è direttamente discendente dalla Costituzione. Ora, signor Presidente, noi possiamo fare tutto, ma prima ancora di farlo e in maniera assolutamente subordinata, essendo d'accordo con quanto detto dal senatore Palma poc'anzi (cioè che questo fosse quantomeno chiarito e introdotto alla Giunta per il Regolamento), avrei gradito - mi scusi, leviamo

Altrimenti, a questo punto, noi introduciamo la fattispecie dell'integrazione dei pareri. Lei capisce bene cosa significa: ogni volta arriva un parere della Commissione bilancio, noi votiamo e alla fine ci accorgiamo che c'è un errore, che non è a questo punto della spalmatura su un triennio; è una inosservanza rispetto alla legge di contabilità, e non è soltanto un'inosservanza teorica, bensì pratica: senza questo chiarimento, nel fare la legge di bilancio del prossimo anno, quanto si andava ad iscrivere

come si farebbe a stabilire? Lo dovrebbe stabilire la Presidenza, ma sulla base di cosa? Sulla base del buon senso? Ecco perché diciamo che questa deroga è molto forte; troppo forte, ad avviso mio e dei colleghi che mi hanno preceduto, perché sia votata. E ritorno all'ipotesi dell'ordine del giorno. Ma al momento in cui si dovesse votare, che questo non costituisca assolutamente un precedente, perché è un'enorme forzatura - questa questa sì - che non ha precedente nella storia di quest'Aula del Parlamento.

ovviamente sulla base della dichiarazione di ammissibilità della proposta emendativa dei relatori sulla ripartizione dello stanziamento annuale, all'ammissibilità di tutte le eventuali proposte che andrebbero sostanzialmente a modificare il testo.

però mi corre l'obbligo di utilizzare anche il paragone che ha segnalato il senatore Palma per avere per avere un metro di valutazione e di misurazione dell'onestà intellettuale di ciascuno di noi. Il provvedimento sulla graduazione degli abbattimenti era a me molte caro perché interessava specificamente gente del mio territorio, e mi rivolsi al senatore Azzollini, esperto di bilancio dello Stato, chiedendogli se quella correzione, ovvero eliminare il 2016 ed inserire nel fondo triennale

di opinioni. Il senatore Azzollini continua, correttamente, con la sua tesi per quanto riguarda l'emendamento dei relatori. Il senatore Tonini ha cambiato opinione e afferma che quell'emendamento può essere di coordinamento perché, pur incidendo sul bilancio annuale, comunque non sposta il fondo che, anche in quel caso, non differenziava nello stanziamento del fondo.

Seguono, nella sostanza dell'*iter*, il medesimo percorso, signor Presidente. Vengono votati, come vengono votati gli emendamenti. Per questo, probabilmente, c'è la confusione dei due termini. Ne abbiamo presentati cinque, come abbiamo presentato cinque proposte emendative semplicemente per un fine estetico, per esaltare la contraddizione in cui è incorsa

registrato in termini chiari è la differenza di comportamento sotto il profilo culturale

va alle Sezioni unite. Ora, mi sembra che il contrasto interpretativo su questo punto sia evidente perché, se per quell'emendamento pochi giorni fa si è deciso che non era sufficiente una proposta emendativa, ma occorreva un emendamento, oggi - per carità, legittimamente - si cambia opinione. Cosa si fa, quando ci sono due opinioni contrastanti? Si va a chiedere all'organo supremo, in questo caso la Giunta per il Regolamento. Signor Presidente, la la Presidenza dovrebbe, correttamente, rimettere alla Giunta per il Regolamento la questione, perché dica se questi emendamenti rientrano nella previsione del Regolamento come proposte emendative o Per questa ragione, io insisto su questa richiesta e le chiedo di fare in modo che l'organo

perché non si è avvalso della consulenza del senatore Azzollini per presentare un emendamento con la ripartizione annuale anziché lasciarla con 20 milioni su base

spesa di 20 milioni in 7, 7 e 6 è una divisione opinabile tanto quanto le altre: io ho proposto 8, 8 e 4, altri hanno proposto 5, 5 e 10 e così via. Il fatto che sia opinabile dimostra che non è un coordinamento, che dovrebbe essere una proposta sulla quale sostanzialmente si converge tutti a livello di logica; in questo caso è una decisione diversa. Non si può stabilire per coordinamento che nel 2017 o nel 2018 si spende un milioni di più o un milione di meno. Se è così, vanno a monte una serie di norme stabilite dalla legge di bilancio e così via.

- con il dubbio che si tratti di un vero coordinamento. In realtà, ritenevamo che non si trattasse di un coordinamento per cui eravamo pronti ad accettare Grazie

l'altro sta osservando il presidente Latorre che sta parlando con un collega, per cui, siccome i relatori neppure ascoltano gli interventi, è normale. *(Commenti del senatore Lumia)*. Bene, visto che adesso mi ascoltano, vorrei ricordare che sarebbe bene che i relatori facessero capire all'Assemblea le cose che propongono, in particolare le proposte di coordinamento.

contrario o favorevole non spiegano il perché, non spiegandone le ragioni, io non lo posso capire, a meno che non sia così chiaro. La proposta di coordinamento per quanto riguarda l'articolo 34 propone sostanzialmente di sopprimere all'articolo 34 il riferimento

si applicano nei procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia già stata formulata proposta di applicazione della misura di prevenzione». Non si tratta di un coordinamento: vuol dire che in questo testo, peraltro approvato dall'Assemblea secondo tutti i crismi della regolarità, si è stabilito che i commi 2-*bis* e 2-*ter* si applicano a taluni provvedimenti.

che, senza coordinamento, si sarebbero svolti secondo una determinata procedura, con tutte le modifiche tecniche previste da questo provvedimento che stiamo esaminando, mentre con il coordinamento non si applicano più e si applicano delle procedure diverse. Poiché questi procedimenti si svolgono

E leggendo il testo io non trovo alcun elemento che spieghi perché, in sede di coordinamento formale, dobbiamo cambiare in modo sostanziale e tutt'altro che formale una norma che è già stata approvata e tra l'altro è stata approvata anche dalla Camera. È vero, per carità, che possiamo cambiare qualunque norma sia stata già approvata dalla Camera, ma questa mi sembra tutt'altro che una modifica di coordinamento.

le questioni regolamentari sono state, a mio avviso, espresse compiutamente dal senatore Palma, io affronterò il problema che abbiamo davanti esclusivamente e sempre dal punto di vista

mi occuperò anche di alcune cose concrete delle quali lei si è occupato poco fa (e mi pare giusto, come sempre, dare risposte puntuali alle sue osservazioni), voglio

Se all'articolo 12 per esempio fosse scritto che si dà un'agevolazione a tutti coloro che hanno gli occhi celesti e in un altro articolo si desse la stessa agevolazione a coloro che non hanno gli occhi celesti sarebbe palese che si tratta di inconciliabilità. In questo caso, non c'è alcun concetto oppositivo, ma soltanto un concetto integrativo: c'è una norma alla quale manca un pezzo, la modulazione annuale dell'onere, e bisogna integrarla. Non devo certamente spiegare a lei la notevolissima differenza esistente tra il concetto oppositivo e quello integrativo. Dunque, noi siamo di fronte a una norma che, così come è, non ha alcun profilo regolamentare; ha un profilo, invece, di sostanza: la mancata aderenza a una norma, peraltro, di diretta derivazione costituzionale, che è quella del principio di annualità del bilancio. Ed è questa. Dunque,

riapprovarlo e le conseguenze sono che la norma è approvata. Quindi, non c'è alcun concetto di inconciliabilità; vi è un problema di integrazione per una norma di diretta derivazione costituzionale; tale norma potrebbe essere superata, ma, si capisce, a prezzo di un *vulnus* notevole, giustificato da motivi che solo il Governo può esplicitare; pertanto il Parlamento oggi si trova di fronte a questa situazione. Cosa c'entri l'articolo 103 del Regolamento onestamente non riesco a capirlo. Ma attenzione, signor Presidente, questa questione (cioè che si tratta di una norma integrativa) è stata palesemente espressa, a mio avviso in modo perfetto, dal Presidente della Commissione bilancio,

dell'emendamento o del subemendamento che la Commissione di merito approva prima dell'emendamento, così che l'emendamento viene parere della Commissione *ex* articolo 81. Si tratta di un emendamento, non c'è altra natura. Che c'entra il coordinamento con l'emendamento? È chiarissimo dal dibattito di quest'Assemblea che si tratta di un emendamento. Su questo emendamento sorge un ulteriore problema, dal mio punto di vista. Oggi si parla di varie modulazioni. A mio avviso, essendo irricevibile il coordinamento su questo punto, sono irricevibili anche le proposte di modifica. È chiaro che i senatori le hanno presentate perché c'è un coordinamento e ritengono di modificarlo.

Tutto era possibile, ma ho avuto la sensazione, signor Presidente, che invece vi sia stata una sorta di ostinazione politica a non vedere una questione che, come al solito, è stata presa più come ostacolo procedurale che come tentativo di collaborare,

la prego, signor Presidente, non introduciamo questo principio. Si faccia un ordine del giorno: la legge, così com'è, è perfettamente aderente al dettato di normazione,

proposta di coordinamento e conseguentemente tutte le altre; chiedere ai relatori che si faccia un ordine del giorno dicendo che bisogna modulare l'ordine; il Tesoro scriva nella relazione di accompagnamento che c'è questo problema e il tutto sarà risolto in perfetta adesione alla sostanza delle questioni. Altrimenti la Costituzione, che prima era troppo

che sono venuti sommessamente, uno dal presidente Ferrara e l'altro dal presidente Azzollini. Da una parte, scrivere che tutto ciò non costituisce precedente, dall'altra, fare un ordine del giorno esplicativo che consenta all'altro ramo del Parlamento di sanare la situazione. di intervenire in questa sede su un dato sostanziale, e anche questo non deve costituire precedente. Lei sa che d'estate si dorme poco, magari ci si riaddormenta alle sette e non si fa in tempo a leggere i giornali. sono così riuscito oggi a compulsare la rassegna stampa prima di arrivare in Aula. Sono stato molto incuriosito dagli interventi dei colleghi Gasparri e Bonfrisco, che hanno fatto riferimento all'articolo di Liana Milella

Il collega Mirabelli ha detto che nessuno aveva presentato emendamenti sugli aspetti che sono stati poi criticati ed è stato puntualmente smentito. In altri tempi

Ieri abbiamo sentito dire dalla bocca dei relatori, del presidente D'Ascola e di molti colleghi della maggioranza, assolutamente uomini d'onore, che in realtà dubbi che hanno una valenza istituzionale (perché non sono dubbi di commentatori, ma sono provenuti dal capo dell'*Authority* anticorruzione, dal presidente della Corte di cassazione e da altri) sarebbero stati formulati troppo tardi

il 20 aprile è stata consegnata una relazione nella quale tutti i dubbi che sono stati esternati negli ultimi giorni erano già evidenti. Chiedo al presidente della Commissione giustizia D'Ascola e ai colleghi relatori, che sono uomini d'onore, erano al corrente di questa relazione e perché il Parlamento non è stato portato a conoscenza di questa relazione per poter intervenire presto.

perché i suoi non l'avevano portato a conoscenza che questo parere era stato messo per iscritto, ripeto, signor Presidente, il 20 aprile. Come è possibile una cosa del genere? Come è possibile che all'interno di un Ministero, non del parere dal magistrato Cantone, che francamente di pareri ne ha dati anche troppi (e spero che questo dibattito sia stato anche un vaccino rispetto agli eccessivi pareri dati da Cantone, che si è espresso persino sulla formazione del Napoli: oggi, come tifoso del Napoli, mi

Anche in quella sede ha affermato, correttamente, che le proposte di coordinamento approvate in Commissione, pur essendo volte ad adeguare il testo alle condizioni poste dalla Commissione recano modifiche di carattere sostanziale, che avrebbero dovuto essere più opportunamente introdotte attraverso la presentazione di veri e propri emendamenti. Che siano modifiche di carattere sostanziale, signor Presidente, lo ha richiamato il senatore

a qualsiasi richiesta di sottoporre una questione alla Giunta per il Regolamento, tranne l'occasione in cui si sarebbe dovuto modificare il sistema di voto per il caso Berlusconi,

si configura come più flessibile e meno formalizzato rispetto alle regole della discussione in Assemblea», mi dico che finalmente abbiamo fatto chiarezza e che in Assemblea queste cose non si verificheranno mai più.

non lo rimettiamo alla Giunta per il Regolamento, a quel punto abbiamo presentato degli emendamenti correttivi di questo emendamento di coordinamento, che tale non è.

norme, che però a un certo punto si sedimentano e trovano un'interpretazione coerente da parte della Corte di cassazione. Pertanto, ciascun giudice, nel valutare l'insegnamento della Corte di cassazione, si può discostare solo se dà un'interpretazione diversa.

non è una risposta a quanto lei ha detto, però rilevo che i presupposti di ogni decisione devono prendere atto delle varie situazioni. Una cosa è la Commissione che dà possibilità all'Assemblea di intervenire,

Signor Presidente, vorrei un attimo ripercorre la vicenda di questo benedetto emendamento, perché forse non è risultato non è risultato così chiaro che l'errore iniziale non parte dalla Commissione giustizia. La Commissione bilancio formula un parere non ostativo «a condizione che». Nelle condizioni - parliamo quindi di una cosa obbligatoria

Mi torna in mente l'articolo 40 del Regolamento laddove, al comma 5, si dice che l'eventuale opposizione deve essere motivata dalla: «insufficienza delle corrispettive quantificazioni», «la verifica delle idoneità della copertura finanziaria ai fini dell'espressione del parere di cui al comma 5, deve riferirsi alla quantificazione degli oneri recati da ciascuna disposizione e agli oneri ricadenti su ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale in vigore.». Evidentemente, così com'è stata formulata la condizione da parte della Commissione bilancio, non risulta conforme a quanto previsto dal Regolamento e conseguentemente dall'articolo 81. Al punto che il presidente Tonini dice che la 5a Commissione si è riunita e ha preso in esame il problema posto dal senatore Azzollini, che l'evidenza dimostrava essere un problema fondato, posto che la norma, votata per errore dalla 5a Commissione,

la Commissione programmazione economica e bilancio, ad integrazione del parere espresso sul testo, conferma il parere non ostativo, e quindi continuerebbe ad attribuirgli una copertura regolamentare *ex* articolo 81, 81, ad una condizione. È evidente, quindi, non avendo ancora osservato e dato seguito a tale osservazione, che poi si è tradotta in una norma di coordinamento, che l'articolo 32 - che ricordo abbiamo votato due volte

questo, Presidente, perché invece che rincorrere norme di coordinamento che, secondo me, con l'articolo 103 francamente non centrano assolutamente nulla,

in buona fede, non sapendo che c'era un problema *ex* articolo 81 rispetto al voto espresso, non capisco perché non si possa dire che vi è stata una irregolarità nel voto. Si torna a votare l'articolo 32 nel testo integrato con la norma di coordinamento e tutti vissero felici e contenti. *(Applausi dei

che il parere della Commissione bilancio è una integrazione del parere stesso sul testo ed è una conferma del parere non ostativo con la seguente condizione e cioè che deve intendersi una specificazione di quello che era già contenuto

pertanto la votazione dell'articolo 32 era irregolare e dovrebbe essere ripetuta.

Grazie

Uno dei motivi per cui ho presentato una proposta di coordinamento è proprio per dimostrare (sicuramente non ha lei, signor Presidente, perché vista la sua perizia non le sfuggirà questo dato) quanto di sostanziale vi sia

ci rendiamo conto, proprio dai contenuti spesi nel testo, che si tratta di emendamenti: la formula è innovativa, è modificativa, le assicuro, signor Presidente, che ho cercato con assoluta sincerità e onestà intellettuale di confrontarmi su questo contenuto e di capire, soprattutto relativamente all'articolo 34, quale sarebbe stato l'esito finale contenutistico, testuale e quindi di merito applicativo,

da loro stessi (posto che, come tutti sappiamo, solo i relatori possono fino all'ultimo secondo presentare emendamenti sul testo all'attenzione dell'Assemblea), ma è stato difficile anche ai

Noi stiamo parlando di un testo che impatterà fortemente sull'assetto legislativo, ordinamentale, giurisdizionale, cautelare, prevenzionale del nostro Paese; un testo destinato ad avere effetti dirompenti, su cui si sono misurati i principali giuristi del nostro Paese del nostro Paese e presidenti emeriti della Corte costituzionale, come abbiamo già detto. Signor Presidente, tutto questo attiene al coordinamento formale del testo. il ministro Orlando presente in quest'Aula. il presidente Cantone ha inviato al ministro Orlando una relazione illustrativa del testo che stiamo per approvare, con un coordinamento finto formale,

Noi stiamo illustrando un testo, come le ho detto, che ha subito in quest'Aula delle mutazioni genetiche assolutamente irregolari. come altri colleghi che già prima di me hanno avanzato questa istanza, sono membro componente della Giunta per il Regolamento, organo tecnico-giuridico caduto in questa legislatura in desuetudine. Presidente, quante volte l'abbiamo pregata, dall'alto della sua corretta e coerente gestione dell'Aula e di tutto ciò che all'Aula è connesso, compresa l'interpretazione del Regolamento, che muove le azioni di tutti noi, di convocare la Giunta per il Regolamento, l'unica in grado di risolvere il problema che ci sta tenendo tutti oggi in quest'Aula? Se noi continuiamo a discutere, signor Presidente, non è perché siamo opposizione brutta, sporca e cattiva, ma perché abbiamo un problema,

evocava una sua interpretazione coerente e immutabile del Regolamento. Signor Presidente, lei e la Giunta per il Regolamento - non ho bisogno di dirlo a lei - svolgete due funzioni diverse. La sua interpretazione coerente e immutabile, come la definisce il senatore Caliendo, non può essere sostitutiva dell'attività della Giunta per il Regolamento; altrimenti per quale per quale motivo esisterebbe la Giunta per il Regolamento, se la sua interpretazione coerente e immutabile potesse tenere luogo della stessa?

Presidente, lei è particolarmente intuitivo e l'ha capito da subito, alle prime due parole. Però io vorrei che chi meno di lei è in grado di interpretare il mio pensiero lo capisse compiutamente. Molto semplicemente, signor Presidente, la prego, questa volta ci ascolti. Lo dirò molto semplicemente, con parole mie. Visto che oggi in quest'Aula si è manifestato un malessere forte su un provvedimento importante, destinato a produrre effetti cospicui, rilevanti ed eclatanti sul nostro ordinamento, non segua la tradizione che ella stessa ha instaurato di non convocare la Giunta per il Regolamento. La convochi

a un'espressione che è stata usata più volte in ogni intervento: «coordinamento formale». Esso prevede diverse tipologie di intervento sul testo prima del voto finale: «correzioni di forma», «modificazioni di coordinamento», rimedi rispetto a «disposizioni già approvate che sembrino in contrasto tra loro», nonché a disposizioni «inconciliabili con lo scopo della legge». Quindi, anche alla luce di una costante prassi applicativa, non vi è alcun dubbio sul significato dell'articolo 103 del Regolamento come norma di chiusura dotata di un sufficiente grado di elasticità al fine di dare coerenza al testo della legge. Siamo arrivati a un punto in cui è necessaria,

ad essa sottoposte dal Presidente del Senato». L'interpretazione del Regolamento si riferisce a tutto, anche all'articolo 103. Se lei non vuole convocarla, dica che non vuole convocare la Giunta per il Regolamento e se ne assume la responsabilità.

1225, 1366, 1431, 1687, 1690, 1957, 2060 e 2089.

affrontando, quest'Assemblea deve dedicare un momento per il ricordo e rendere omaggio a un grandissimo artista, attore di cinema e televisione, scrittore e sceneggiatore che ci ha appena lasciati, Paolo Villaggio.

e tutte le onorificenze che ha ricevuto durante la sua lunghissima carriera. In fondo poi lo conosciamo bene tutti, lo citiamo, lo vediamo ancora aggirarsi tra noi, perché nel suo genio ha descritto noi italiani come pochi altri hanno saputo fare. Ultraitaliano, come lo ha definito sul *blog* Beppe: mi pare un aggettivo perfetto. Sì, perché coi suoi personaggi e la sua poetica è stato spietato nel mostrarci come siamo veramente, grottesco se volete, surreale ma pregnante e denso di realismo. Tanto è vero che continueremo a citarlo per sempre, perché con i suoi personaggi, più di tutti ha centrato in pieno chi siamo, con i nostri difetti e le nostre piccolezze d'animo, senza mai senza mai assolverci, senza mai falso buonismo. E ha saputo descrivere quanto possa essere dura, ma anche dolce, la realtà di chi tutti i giorni affronta la vita, magari con una marcia in meno ma con un cuore grande, apre una nuova finestra") **(ore 13,09)** (Segue AIROLA). L'insegnamento più bello sta proprio in quei pochi ma fantastici momenti di rivalsa del suo personaggio più famoso, che ci hanno commosso quasi fino alle lacrime per la gioia, come per la famosa battuta alla proiezione del *super* megadirettore malato di cinema d'*essai* o per il sasso tirato alle finestre dell'ufficio dove lavorava dicendo la famosa battuta «Mi avete fregato tutta la vita». Consapevolezza che mi auguro ci accompagni per sempre. *((Applausi dal Gruppo M5S)*. Caro Paolo Villaggio, non ti dimenticheremo mai. Sono certo che il tuo messaggio, i tuoi personaggi, la rappresentazione della natura umana e culturale italiana ci resteranno nella mente e nel cuore per sempre, perché sei riuscito a toccarci nel nel profondo dell'animo. Grazie Paolo! Grazie

per tante difficoltà, ma certamente uno dei motivi più importanti è legato alla straordinaria sordità di un direttore generale che guida quella direzione e che, chiuso nella sua torre eburnea, ha ridotto - fino ad azzerare praticamente al minimo - ogni rapporto e forma di dialogo con il personale sanitario dell'azienda, con conseguenze facilmente immaginabili sulla salute delle cittadine e dei cittadini di tutta la comunità iblea. Intervengo in Aula questa mattina perché in questi giorni davvero la misura è colma. Infatti, in quella Provincia, da un punto di vista sanitario, regnano l'ansia, la preoccupazione, la confusione legata al trasferimento dal vecchio ospedale a quello nuovo. Per chi non conosce questa storia,

Capite bene che le scadenze e gli obiettivi sono molto importanti, per tanti motivi. Ebbene, è stato deciso un trasferimento da un ospedale all'altro quando ancora quello nuovo non era assolutamente adeguato da un punto di vista funzionale. C'è stata fretta, frenesia di andare per far vedere che si manteneva un impegno. È onorevole che si mantengano gli impegni, ma bisogna che gli ospedali siano adeguati e funzionanti perché lì si curano le acuzie e le persone che stanno male vanno sostenute nella maniera più importante, più giusta, più corretta e più professionale possibile. Bene, è successo che, purtroppo, l'ospedale nuovo non era adeguato; la procura ha messo i sigilli alle sale operatorie e così siamo arrivati a un risultato davvero drammatico, per cui il vecchio ospedale non è più agibile perché sono state dismesse le sale operatorie e trasferite

sono oberate, sono già piene dei loro pazienti, sono sovraccaricate, non hanno personale sufficiente e si chiede ai medici e al personale di sovraccaricarsi di tutto quello che faceva l'altro ospedale. Questo non è possibile perché non ci sono né i posti letto né il personale. Siamo nel periodo estivo, quindi il personale dovrebbe andare in ferie; sappiamo che ha bisogno di turni di riposo perché non può essere sovraccaricato e allora c'è la paralisi totale. C'è uno sforzo enorme da parte di tutto il personale che si mette a disposizione, ma c'è l'incapacità di gestire questo momento di confusione che, ad oggi - ringraziando Iddio - non ha determinato conseguenze gravi; ma non sappiamo che cosa potrà accadere nei prossimi giorni.

Chiedo che si rimuova il direttore generale, perché in questo momento non ha più la lucidità e la serenità per guidare una realtà davvero in grande sofferenza. Siamo in estate, aumenta la presenza delle persone in quella zona, quella di Montalbano

in dovere, da cittadina, da rappresentante istituzionale, da medico, di dire queste cose ad alta voce perché non voglio essere corresponsabile. Lo ripeto da anni ma adesso davvero la misura è colma. 4 luglio 2017, ore 20,40 di un'altra giornata superata nonostante le difficoltà quotidiane affrontate silenziosamente da tutta l'umanità: proprio nel momento della quiete familiare, mortai e lanciagranate hanno colpito subdolamente un villaggio del distretto Füzuli dell'Azerbaigian distruggendo per sempre due vite e rinnovando il terrore in una comunità alla sola ricerca di pace e progresso, Chi ha avuto l'ardire di uccidere una nonna e la sua nipotina di due anni e ferire gravemente altre due persone sono le forze armate armene, incuranti della visita dei co-presidenti del gruppo di Minsk dell'OSCE nella regione e dei relativi inviti al cambiamento dello *status quo* di occupazione tramite negoziati sostanziali e seri. L'Armenia sta conducendo attacchi sistematici, deliberati e mirati alla popolazione civile specialmente contro donne, bambini e anziani. I video di questi attacchi sono in rete in tutto il mondo; sono attacchi diretti e deliberati, quasi attentati terroristici, contro la popolazione civile azerbaigiana e costituiscono una grave violazione del diritto internazionale umanitario e dei diritti umani, della Convenzione di Ginevra del 1949, della Convenzione sui diritti del fanciullo e della Convenzione per la Esistono, come se non bastasse, molte risoluzioni internazionali, comprese quattro risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che impongono il ritiro dell'Armenia dai territori occupati dell'Azerbaigian e il ritorno dei profughi azerbaigiani (circa un milione di persone) alle loro terre. Tali documenti vengono costantemente ignorati, dimostrando come l'obiettivo di Yerevan coincida con il mantenimento dello *status quo*, con provocazioni sistematiche e sabotaggi lungo la linea di confine. La soluzione del conflitto non può prescindere dal ritiro delle forze armate dell'Armenia dai territori occupati, la cui presenza è il maggiore ostacolo alla soluzione del conflitto. Questa violenza deve essere fermata. Il Governo italiano, in considerazione del suo ruolo alla presidenza OSCE nel prossimo anno, e di membro della *troika* dell'OSCE, è chiamato a lavorare in questa direzione, per una soluzione rapida di questo terribile

Il mio Gruppo vuole oggi ricordare gli ottant'anni dalla scomparsa di un nostro collega, perché è stato senatore del Regno dal 30 aprile 1914 al 20 luglio 1937. Sto parlando di Guglielmo Marconi.

perché è un collega, ma perché chi vi parla abita una zona cara al senatore Marconi, il nostro primo premio Nobel per la fisica del 1909, che ha dato lustro all'Italia nel mondo: a lui sono intitolate strade, golfi, punti storici (io ne ho visitato uno in Canada, dove ha fatto un famoso esperimento).

comunicazioni con la telegrafia senza fili, tramite onde radio e il radiotelegrafo, che sono stati sistemi che hanno dato il alle radiotelecomunicazioni e alla televisione. Lo ricordo in un'immagine televisiva - ci sono ancora, se Dio vuole, dei programmi a lui dedicati - quando con Pio XI ha fondato «Radio Vaticana»: ha fatto parlare per la prima volta il Papa e l'hanno potuto sentire in tutto il mondo contemporaneamente. Era un nostro collega, ricorrono ora gli ottant'anni dalla sua

autodidatta, non in un garage ma in una stanza vicino a casa, in una notte di dicembre ha svegliato papà e mamma

alla figlia Elettra, che porta ovviamente il nome di un'importante nave su cui sono avvenuti gli esperimenti. Ricordo anche anche i superstiti del Titanic, del più grosso disastro che ha avuto una nave: centinaia sono stati salvati grazie al fatto che, con l'SOS, si

la loro sopravvivenza si deve a lui. Signor Presidente, il Gruppo rivolge un saluto affettuoso alla figlia e ai familiari di questo nostro collega collega senatore, che ha dato lustro all'Italia con un premio Nobel vero, partendo come autodidatta. Aveva ragione qualcuno quando diceva che effettivamente siamo

le loro preoccupazioni e gli impegni che erano stati assunti nell'8ª Commissione del Senato, attraverso il presidente Matteoli e il sottoscritto, hanno trovato una

In particolare, viene garantito il trasferimento di tutti i lavoratori, esclusi i dirigenti; vengono garantiti il trascinamento e la conservazione di tutti i diritti maturati dai lavoratori, a prescindere dallo strumento formale del trasferimento; soprattutto, viene garantita l'applicazione del contratto collettivo nazionale di settore e di quello di secondo livello o territoriale applicato dal soggetto gestore uscente. La seconda modifica, altrettanto importante, contenuta nel secondo emendamento che abbiamo presentato, che ci auguriamo possa essere

dalle norme del trasporto pubblico inserite nella manovrina, passi attraverso il primo utilizzo dei lavoratori non idonei, in modo da evitare qualunque rischio di un loro licenziamento. Mi sembra Mi sembra importante dire da questi scranni del Senato ai lavoratori che oggi hanno scioperato che siamo a un passo dalla soluzione del problema e che l'8ª Commissione del Senato, così come si era impegnata a fare in sede di audizione delle sigle sindacali, ha preso preso atto del lavoro svolto dal tavolo del MIT e l'ha trasformato in un'azione parlamentare. A questo punto, visto che quest'Assemblea voterà a breve tale provvedimento, con l'approvazione di questi due emendamenti saneremo la vicenda che ci ha portato all'abrogazione del regio decreto n. 148 che, come sappiamo molto bene, per i lavoratori del trasporto pubblico locale è sempre stato un punto fermo.

per chiedergli come fosse compatibile la nomina, che abbiamo letto sui giornali, del coordinatore della struttura tecnica di missione del Ministero delle infrastrutture, professor Cascetta,

allora del tutto strano che venisse fatta questa nomina, ma poi ho letto una notizia

perché abbiamo il documento nel quale egli dichiara di essere un professore ordinario, a tempo pieno, presso l'Università Federico II, di Napoli, dalla quale riceve anche un emolumento - che fa il presidente di una concessionaria privata, che è nominato presidente delle Rete autostrade del mare e che, oltretutto, così come riportato nella sua dichiarazione, percepisce un vitalizio in qualità di ex assessore della Regione Campania. Tutto questo non viola alcuna norma, non viola alcuna legge.

Questa normalità è inconcepibile: il nostro Paese è pieno di persone brave e competenti e non è possibile che siano sempre le stesse persone a ricoprire tantissimi incarichi, tutti a carico delle finanze pubbliche. Questo modo di fare è inaccettabile e bisognerebbe che, per una volta, si iniziasse a capire che è necessario mettere in moto le capacità incredibili ed enormi di questo Paese, evitando che i soliti baroni - perché è di loro continuino a fare il bello e il cattivo tempo. L'Italia può farcela se smantelliamo queste cose.